Come comunicato nel corso della seduta antimeridiana, dopo l'intervento del rappresentante del Governo, ciascun Gruppo potrà intervenire per cinque minuti ed il Gruppo Misto per dieci minuti. Ha facoltà di parlare il sottosegretario di Stato per la difesa Forcieri. difesa*. Signor Presidente, onorevoli senatori, un gravissimo lutto ha colpito il Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI) con la perdita del maresciallo capo Lorenzo D'Auria, rimasto gravemente ferito in Afghanistan, spentosi in mattinata presso il Policlinico militare del Celio in Roma. In questa dolorosa e triste circostanza desidero innanzitutto esprimere, a nome del Governo, del Servizio e delle Forze armate, le più sincere e profonde espressioni dì partecipazione e cordoglio alla famiglia del giovane militare. Al Servizio va tutta la nostra solidarietà per l'opera che il personale svolge quotidianamente, anche in difficili momenti come l'attuale, ed in contesti anche molto pericolosi, con professionalità ed abnegazione. Il sottufficiale era un militare inquadrato nel Servizio - al momento ancora denominato Servizio per le informazioni e la sicurezza militare - e, in quanto tale, istituzionalmente preposto a garantire la cornice informativa e di sicurezza necessaria al successo della nostra missione in Afghanistan. Più nel dettaglio, il nostro operatore, unitamente ad un altro sottufficiale, era incaricato di mantenere e sviluppare dei rapporti con la popolazione civile e le autorità locali per individuare le migliori forme di collaborazione e convivenza, nonché di raccogliere informazioni utili a tutelare la protezione del contingente dalla minaccia terroristica. Tale compito, che prevede l'effettuazione di complesse attività al di fuori della cornice di sicurezza garantita dalle nostre unirà militari presenti in teatro, e che quindi implica l'assunzione dei conseguenti rischi, ha consentito nei diversi anni di permanenza in area afgana del contingente, di evitare numerosi attacchi terroristici, non solo alle truppe nazionali, ma a tutta la forza ISAF. Venendo alla descrizione dello specifico evento riguardante il sottufficiale deceduto, desidero richiamare, in questa sede, i principali elementi di informazione che il signor ministro, onorevole Parisi, ha fornito il 24 e il 26 settembre settembre scorso rispettivamente presso l'Aula della Camera dei deputati e la 4a Commissione (Difesa) del Senato della Repubblica. Nel corso di una missione informativa nella provincia di Herat, il maresciallo D'Auria ed un altro militare del Servizio, assieme ad un interprete ed un accompagnatore afgani, sono stati fermati e sequestrati, nella mattinata del 22 settembre, vicino a Shindad, da un gruppo afgano di uomini armati. A seguito del mancato collegamento radio hanno avuto inizio le operazioni di ricerca. Il comandante del *Regional Command West* attuava tutte le predisposizioni necessarie, mettendo in allerta gli assetti disponibili e, in particolare il velivolo *Predator*, la componente elicotteri CH-47 e A-129 Mangusta e le forze ISAF presenti nell'area di operazione, al fine di essere in condizione di fornire con rapidità ogni tipo di sostegno possibile in relazione allo svilupparsi della situazione informativa sulla sorte dei quattro ostaggi. Veniva quindi instaurato uno stretto raccordo con il comandante italiano delle forze speciali ISAF operanti nella regione Ovest, al quale veniva affidata la responsabilità di gestire la situazione e di pianificare, avvalendosi anche di altri assetti alleati disponibili, un eventuale intervento per liberare gli ostaggi ove se ne fossero presentate le condizioni. Pertanto, veniva tenuto in volo con continuità un velivolo senza pilota *Predator* per monitorare l'area di possibile presenza degli ostaggi e venivano ridislocati nella base di Farah assetti elicotteristici nazionali ed alleati. Nel frattempo, col concorso degli elementi informativi messi a disposizione da tutti gli alleati, nonché grazie ad elementi di *intelligence* Humint ottenuti dai nostri Servizi in teatro, si veniva delineando un quadro informativo che individuava, con buone probabilità, la presenza degli ostaggi nella parte meridionale della regione Ovest (distretti di Shindad e Farah). Nel primo pomeriggio del 23 settembre, a seguito della localizzazione dei rapitori e della successiva monitorizzazione dei loro movimenti, le forze ISAF hanno ricevuto dal ministro Parisi, in accordo con il Presidente del Consiglio, con il quale è stato mantenuto durante tutta la vicenda un contatto costante, l'autorizzazione a pianificare ed eventualmente condurre un'operazione militare per la loro liberazione, qualora si fossero presentate le condizioni ambientali necessarie per un positivo intervento. In tale circostanza, sono state impartite direttive chiare ed essenziali. In primo luogo, l'obiettivo di un'eventuale operazione di liberazione doveva tendere alla salvaguardia della vita di tutti e quattro gli uomini rapiti. Si doveva, inoltre, ridurre al massimo il rischio di coinvolgimento di civili afgani. Sulla base di queste indicazioni, l'operazione è, pertanto, materialmente scattata alla prima - e, verosimilmente, ultima - occasione che si è resa disponibile. Avendo localizzato, nelle prime ore della giornata del 24 settembre scorso, due veicoli ruotati correlabili ai rapitori che si dirigevano dalla provincia di Farah verso il Sud dell'Afghanistan, si è deciso di intervenire. L'azione è stata pianificata e condotta insieme da forze speciali ed elicotteri italiani e britannici ed ha portato alla liberazione degli ostaggi. Al pari della copertura informativa assicurata dall'*intelligence*, anche l'azione diretta ha visto il coinvolgimento sia di unità italiane, sia di reparti alleati, tutti facenti parte della missione ISAF. Nell'ambito dell'alleanza, infatti, esistono procedure e meccanismi di coordinamento e di intervento appositamente predisposti per le varie circostanze. Questi meccanismi sono entrati regolarmente in funzione anche in quest'occasione, dimostrando l'assoluta validità operativa della cooperazione fra alleati. L'azione di liberazione è stata purtroppo cruenta, con l'uccisione di otto rapitori, giacché i criminali si sono dimostrati assolutamente risoluti a reagire con le armi fino alle estreme conseguenze. Nel corso dell'azione, risultavano presenti tre prigionieri (due militari del servizio ed un afgano), tutti rimasti feriti. Tutti e tre i rapiti, al momento della liberazione, sono stati trovati ammanettati e bendati in una delle auto con le quali i rapitori stavano fuggendo. Le condizioni del maresciallo D'Auria sono apparse da subito gravissime, tanto da richiedere necessariamente il ricorso ad un respiratore artificiale. Gli altri due feriti non presentavano lesioni di particolare gravità. Successivamente, il giorno 26 settembre, è stato predisposto con un volo il rientro in Italia del maresciallo D'Auria. All'atto del ricovero all'Ospedale del Celio, il sottufficiale si presentava in stato di coma profondo areflessico con assenza di attività respiratoria spontanea, con supporto ventilatorio artificiale. Durante la degenza, è stato costantemente garantito il supporto dei parametri vitali; nel pomeriggio di ieri, si assisteva ad un progressivo deterioramento dei parametri clinici, perdurando l'assistenza farmacologica e meccanica; deterioramento in mattinata ne ha portato al decesso. Nella giornata di domani, venerdì 5 ottobre, verrà eseguita l'autopsia, come disposto dall'autorità inquirente. Oggi, nel concludere, voglio riaffermare che sentiamo ancor di più un grande obbligo di riconoscenza nei confronti dei nostri militari e del personale dei Servizi*. Essi danno prova di straordinaria forza interiore, sopportando grandi sacrifici, sino al contributo delle loro stesse vite. Anche in quest'occasione, sentiamo il dovere di rivolgere loro il nostro commosso pensiero e lo rivolgiamo sapendo che tutta l'Italia si unisce a noi nel dolore e nella gratitudine per il loro sacrificio.

di unirmi personalmente al cordoglio della famiglia D'Auria per la perdita del maresciallo capo Lorenzo e di rendere pubblicamente omaggio a chi serve il Paese in condizioni estreme di pericolo. Mi unisco, per questo, alle parole dei del Governo e del ministro Parisi, che ha espresso profondo dolore per la morte di un uomo generosamente impegnato in una missione di grande valore, di grande valore, al servizio della sicurezza e della pace. Ritengo un dovere istituzionale essere vicino ai suoi cari, riconoscendo l'alto valore di una vita generosamente sacrificata per il bene dell'intero Paese. È un esempio morale di lealtà e altruismo che sento il dovere di onorare con un pensiero di affetto e di profonda riconoscenza. Questo lo faccio anche a nome dell'Udeur e dell'Italia dei Valori.

al dolore della Nazione, anzitutto, per questo caduto che oggi ci troviamo a dover ricordare. Mi permetta di aggiungere solidarietà alla famiglia, a quella splendida compagna che ha voluto unirsi in matrimonio *in* *articulo mortis*, ha voluto cioè dare un senso alla loro vita, e credo che questo sia uno dei gesti più belli che si possano compiere. Signor Sottosegretario, mi scuso per aver ascoltato solo la parte finale del suo intervento, che credo ci sia stato anche qualche elemento di vergogna in questa storia. Questo soldato, rientrato a Roma, non ha trovato uno straccio di autorità ad accoglierlo, come è stato denunciato nell'Aula del Senato; il rimpatrio di quello che possiamo definire un eroe italiano avvenne senza le autorità dello Stato italiano. Credo che questo non sia bello per la nostra Repubblica; spero si tratti di una pagina che sarà possibile rimuovere facendo opere concrete per quanti si battono per la libertà. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi, mi auguro di non assistere più in quest'Aula ad un Parlamento che si divide perché c'è qualcuno che vuole rinunciare ad esprimere abbracci corali ai nostri soldati, a qualunque livello essi siano inquadrati, che vanno in terra straniera per difendere la pace, in missione di pace. Spero che quando si dovrà ridiscutere del rifinanziamento di queste missioni non ci si debba più dividere, che il Parlamento decida finalmente e unitariamente di mandare segnali concreti anche nell'approvazione delle norme al nostro esame, per far sentire a questi soldati che non li ricorderemo solo da morti, ma vogliamo aiutarli finché sono in vita. sostegno pieno, libero, incondizionato alle nostre truppe. Vorrei venisse il momento in cui il Parlamento si decidesse ad esprimersi in libertà contro i tagliagole.

Il secondo pensiero va alla sua famiglia, ai tre piccoli figli, alla moglie, ai genitori. Infine, un pensiero a tutti noi, alla comunità nazionale, a noi che più o meno direttamente abbiamo inviato questo figlio d'Italia in un luogo decisamente difficile. Il sottosegretario Forcieri, nello spiegare le motivazioni di questo suo servizio, ha parlato di garantire la cornice informativa e di sicurezza; un termine certamente tecnico, ma forse un po' riduttivo, perfino nei confronti di quella che in realtà - non solo per il giovane maresciallo D'Auria ed i suoi colleghi, ma per tutti i giovani che oggi sono impegnati su questi fronti - è un po' una missione, non è soltanto un mandato di servizio. È un ruolo per il quale sicuramente i giovani come D'Auria vengono addestrati e anche da D'Auria e dal suo collega ricoperto sicuramente molte altre volte con successo, in missioni più fortunate dalle quali erano rientrati. ad un certo punto, anche le cose più difficili e pericolose possono apparire facili, perfino di *routine*. C'è anche magari, da parte di chi pratica queste delicate professioni, un'assuefazione al rischio e al pericolo. Ecco allora (non è certo né il momento, né il luogo per avviare qualsiasi polemica, né per parlare con accenti che non siano esclusivamente di commozione) che abbiamo il dovere di consegnare non solo al Governo, ma alle nostre coscienze un messaggio, una lezione che può scaturire da un episodio così doloroso. Non è il caso di recriminare su nulla, salvo che sulla perdita di questa vita. Non possiamo però passare sotto silenzio il grido angoscioso non solo di dolore, ma anche di rammarico che i familiari hanno consegnato in questi ultimi giorni ai microfoni e alle pagine dei giornali, con un interrogativo decisamente struggente:

ripeto - dei sentimenti che ci debbono animare in questo momento, non può non colpire chi ha il dovere di organizzare a monte questo tipo di Servizi e di prestazioni. Non è che, magari proprio per abitudine, per il logorio della *routine* quotidiana, si sia sottovalutato un margine di rischio che evidentemente era più grande di quanto fosse previsto? Ecco, allora, che a questo punto le dinamiche e le responsabilità dell'azione passano un po' in secondo piano. Francamente, non mi interessa molto conoscere il nome e il cognome della pallottola o delle pallottole che hanno ucciso il maresciallo D'Auria e che hanno ferito i suoi due compagni di missione. A questo punto non ha alcuna importanza. È un compito, è una preoccupazione che spetta soltanto all'autorità ed alla magistratura militari. Resta la lezione di fondo di questo tipo di presenza degli italiani in luoghi e focolai di guerra e resta, ogni volta che accade qualcosa di irreparabile,

Certo, parole toccanti, ma io sono tra coloro che preferiscono un altro motto: «Beato il popolo che non ha bisogno di eroi», pur comprendendo la necessità, il dovere di celebrarli quando, purtroppo, essi vengono a trovarsi sulla nostra strada.

che in questo momento, nei vari focolai di guerra e nelle turbolenze internazionali, stanno onorando il nostro Paese, correndo gli stessi rischi per i quali molte volte si torna a casa e altre, come nel caso del maresciallo D'Auria, si lascia un vuoto incolmabile.

le parole del sottosegretario Forcieri ci hanno riportato quello che già avevamo sentito nel corso dell'audizione del ministro Parisi, e non poteva essere altrimenti. ha spiegato una dinamica complessa, difficile, che ha portato alla morte del soldato D'Auria.

Quindi, c'è qualcosa di più complesso, che non può essere visto semplicemente come una guerra da fare, punto e basta: c'è una guerra a cui occorre trovare una soluzione politica. Una soluzione, quella della possibilità di superare questo stato di guerra, che può permettere di avere più giovani a casa e meno eroi da ricordare.

e a tutti gli altri giovani soldati italiani che sono ancora lì, probabilmente esposti, ai quali auguriamo di poter rientrare in Patria in un'altra maniera.

Il problema dell'Afghanistan però era diverso da tutti gli altri: erano state infatti annunciate azioni di inasprimento della lotta, della resistenza, sul posto e noi nelle varie sedi chiedemmo al Governo in quali condizioni i nostri militari avrebbero affrontato questo periodo di recrudescenza delle violenze annunciate. Il ministro D'Alema rispose dichiarando, oltre al resto, che non si sarebbe inviato un uomo in più, né un nuovo armamento, né nuove dotazioni. Il punto allora diventava: potevamo noi a cuor leggero rifinanziare, riapprovare, quella missione, conoscendo le condizioni in cui si trovavano i nostri militari? Vero è che in questo caso vi è stato un rapimento, dunque una questione relativamente nuova, ma dipende un po' da tutto un contesto di protezione. A detta del Governo, noi siamo lì per una missione di pace; però è anche vero che quello è un teatro di guerra e questi fatti, purtroppo, lo stanno a dimostrare. Noi dobbiamo rimanere in Afghanistan, perché il primo problema che ha tutto il mondo, tutto l'Occidente è il terrorismo internazionale

I nostri militari devono avere tutto ciò che serve, senza ipocrisia da parte della sinistra, per stare lì e fare il loro lavoro con le garanzie minime di autodifesa e di protezione anche personale. Non è possibile, però (e qui una parola va spesa, anche se il momento non è quello più adatto) che si facciano speculazioni politiche in questi momenti.

i terroristi internazionali sanno perfettamente cosa accade nel nostro Paese, conoscono benissimo Rifondazione Comunista, Caruso e le sue iniziative, sanno perfettamente cosa ha detto Diliberto e sanno anche gli effetti che che producono quelle loro dichiarazioni. Non si può fare sciacallaggio politico sulla pelle dei nostri ragazzi, perché queste dichiarazioni hanno un'eco tale da mettere a repentaglio la sicurezza del nostro Paese e del nostro contingente.

cordoglio e solidarietà, pensando anche ai ragazzi che ancora sono lì, forse non del tutto protetti, e sperando che possano rientrare tutti a casa. *(UDC)*. Signor Presidente, mi unisco al cordoglio per la morte di Lorenzo D'Auria

due mesi. Di fronte a questo evento tutti noi siamo tentati, vivendo in una sede politica che ha visto grandi passioni intorno a questo intervento delle forze NATO in Afghanistan,

Credo però sia il caso, almeno di fronte a questa bara, di fermare e calmare le nostre passioni. Avremo modo di tornare a discutere di tale questione, ma mi fermerei mi fermerei qui, perché questo giovane Lorenzo è uno dei tanti figli migliori di questa nostra Italia, Italia, fa parte di tutti coloro che sono morti per la difesa della nostra identità nazionale, del nostro Stato. Il mio pensiero va ai nostri morti di Nasiriya, ai caduti delle forze dell'ordine, della magistratura, di uomini del servizio civile che in qualche modo hanno voluto rendere un servizio alla comunità nazionale. C'è una Italia

Paese, ma c'è un'altra Italia che tutto questo tutela e favorisce. La nostra attenzione non può non andare, con tutto il rispetto, a questa Italia: l'Italia dei doveri che non si antepone all'Italia dei diritti; anzi, è l'Italia che garantisce i diritti, perché non c'è un'Italia dei diritti se non c'è un'Italia dei doveri, non c'è una comunità internazionale dei diritti se non c'è una comunità internazionale dei doveri.

in Italia, come quelli americani, dove sono sepolti tanti giovani che vennero in quegli anni, lontani dalla loro patria a liberare questo Paese non come invasori, ma unendosi alle forze che amavano la libertà in questo Paese. Allora riesco a pensare al sacrificio di questo giovane in Afghanistan in questa cornice che in quegli anni animò tanti giovani in Italia per la conquista della libertà. Ecco, questi sono i giovani italiani che ripagano la comunità internazionale stando vicino a migliaia di giovani, uomini e donne in Afghanistan, che hanno fatto la fila per votare e per avere uno Stato libero. Solo così riesco a capire questa morte. Diversamente

Presidente, Sottosegretario, colleghi, il 13 settembre, due giorni dopo l'attentato alle Torri gemelle, un'associazione di donne, di cui faccio parte, emise il seguente comunicato: guerra di ritorsione o di aggressione e terrorismo sono parimenti crimini contro l'umanità. Essi non si elidono ma si fomentano. Pensare di spegnere il terrorismo con la guerra è come credere di spegnere un incendio con la benzina. Per questa ragione, la nostra posizione sul terrorismo è che non la si sconfigge con la guerra; opinione probabilmente ormai provata. Ringrazio il sottosegretario Forcieri per aver dato del tragico evento una ricostruzione molto politicamente corretta, tenendo conto e dimostrando, salvo eventuali esiti contrari delle inchieste, che il nostro contingente si attiene rigorosamente alle regole di ingaggio che ha avuto. E di questo volentieri gli do atto. È molto importante che non si scivoli insensibilmente verso dei coinvolgimenti che il Parlamento non ha approvato. Parlamento non ha approvato. Voglio ancora dire, però, che nella sua esposizione una cosa mi ha colpito: ci fu un consenso dato dal Ministro della difesa, insieme al Presidente del Consiglio, all'operazione militare per la liberazione. Non è stato coinvolto per niente il Ministero degli esteri? Non si è mai pensato di avere dei contingenti misti, militari-diplomatici, per queste operazioni?

varie forme di intervento e, del resto, sappiamo che ogni qualvolta un esercito regolare ne incontra un altro, chi viene catturato si chiama prigioniero di guerra ed ha delle sue tutele di diritto internazionale.

catturavamo qualche soldato nazista per ottenere lo scambio con dei partigiani prigionieri. È normale in tutte le situazioni in cui c'è esercito regolare ed ambiente di guerriglia. In queste tragiche vicende ci sono sempre anche delle bande di predoni; nel qual caso si tratta di sequestro di persona a puro scopo di vendita di carne umana. Abbiamo ormai una tipologia significativa di tutti questi eventi. Quindi dovremmo, secondo me, avere una composita preparazione

La vicenda che ci è stata presentata ha carattere di particolare tragicità per la giovane età di chi è rimasto poi vittima e anche per alcune vicende. Voglio qui sottolineare,

Non sempre è possibile il matrimonio *in* *articulo* *mortis*: quando si muore all'improvviso non è possibile. Lo Stato italiano, che accetta che la Chiesa intervenga *in* *articulo mortis,* di suo non riconosce

essere la vedova del maresciallo D'Auria, ma ancora di più essere la vedova del carabiniere che non poté nemmeno partecipare ai suoi funerali. Mi chiedo allora se, indipendentemente dalle espressioni

parlo a nome del Gruppo di Alleanza Nazionale, ma, se mi è consentito, anche come vecchio direttore dei Servizi. Non risponderò o non commenterò l'intervento del Sottosegretario, anche perché egli ha fedelmente ripetuto quello che già il Ministro ci ha detto in Commissione, comunque, in quell'occasione, AN ha espresso la sua solidarietà e la sua approvazione per come il ministro Parisi e i suoi collaboratori hanno gestito il discorso relativo alla cattura e poi alla liberazione con il cuore pieno di tristezza. In questo momento uno si sente veramente piccolo, come credo vi sentiate tutti voi: un senso di impotenza, non si può fare nulla. Il maresciallo D'Auria è caduto in servizio; è stato rapito e poi, nel momento della liberazione, è stato ferito gravemente. Abbiamo sperato, credo tutti, Abbiamo sperato, credo tutti, nonostante le notizie, che il maresciallo potesse salvarsi, ma così non è stato. Il maresciallo è caduto, come si dice, nell'adempimento del suo dovere, in una missione che si chiama di pace, ma che io chiamerei, come tutte le altre, di aiuto a quei popoli.

tutti coloro, militari o non militari, che accorrono in aiuto delle popolazioni meno fortunate della nostra, può essere più comprensibile. in una missione di aiuto, facendo il proprio dovere, come hanno fatto finora e fanno sempre i nostri soldati, rischiando la loro vita e, a maggior ragione, gli appartenenti ai Servizi segreti. appartenenti ai Servizi segreti si sacrificano coscientemente. Non c'è nessuno che entri nei Servizi segreti e svolga missioni di carattere operativo che metta in discussione il fatto che può rischiare la vita. Quindi, è un sacrificio cosciente del quale tutti noi dobbiamo renderci conto. La nostra solidarietà va certamente alla famiglia, commossi anche per questo meraviglioso episodio del matrimonio quasi nel momento della morte. Il pensiero del Senato va certamente a tutti gli altri

in questi momenti si vive una partecipazione autentica, si rivedono anni e anni di attività, di servizio. Poi, in questo momento, come qualcuno ha detto in precedenza, la gioia anche di sentire una partecipazione corale, che eleva certamente il tono di certe situazioni che si verificano dentro quest'Aula in altre occasioni. Onore, quindi, a questo soldato italiano che certamente ha illustrato la frase: «morire per la Patria».

tutta la solidarietà del Gruppo di Forza Italia ai familiari alla giovane sposa che *in articulo mortis* si è sacramentalmente e civilmente accompagnata al marito. È difficile prendere la parola in una circostanza come questa per dire cose non banali che abbiano riferimento non soltanto alla solidarietà, ma anche all'impegno che i nostri militari stanno svolgendo in Afghanistan. In quel Paese ci siamo perché il Governo legittimo dell'Afghanistan ci chiede aiuto collaborazione anche militare per poter instaurare la democrazia e la pace contro il terrorismo di matrice talebana. inoltre, perché l'Alleanza atlantica e l'Unione Europea, con tutti i suoi Paesi fondatori, sono presenti in quest'opera che è insieme politica e militare. A partire da domani, insieme con altri colleghi, sarò all'Assemblea parlamentare dell'Alleanza Atlantica nella sede in cui si discuterà del bilancio, ma anche delle prospettive della missione in Afghanistan, che è definita dal suo segretario generale come la più importante missione militare che, per la riconquista della pace o per il suo consolidamento, abbia fatto l'Alleanza atlantica. Noi abbiamo assunto questa responsabilità. Il Governo attuale ha raccolto il seguito di questa responsabilità - ripeto - orientata a dare pace con tutti gli strumenti possibili quando si tratta di avere contro un nemico che usa l'arma più insidiosa che è quella terroristica.

che abbiamo allegato alla nostra partecipazione a questa missione. Lo ha detto con molta forza l'ex ministro degli affari esteri e vice presidente del Consiglio Gianfranco Fini, parlando di questo gravissimo incidente che è capitato al nostro contingente, nel momento in cui ne abbiamo avuto notizia.

Se quel Paese, anziché chiederci aiuti militari, ci chiede un aiuto di carattere diplomatico, il nostro Ministro degli esteri si è dichiarato disponibile

a meno che non lo facciamo in sede NATO, per trattare con coloro che sono considerati ancora i nostri nemici combattenti e che uccidono i nostri militari. Ecco la ragione per la quale credo che, al prossimo rinnovo dell'impegno finanziario, noi - io senz'altro lo farò - porremo il tema del rafforzamento della nostra posizione.

Non si può sfuggire da questo dilemma: o si rafforza il nostro contingente in rapporto a ciò che l'Alleanza atlantica ci chiede, oppure, francamente, l'altra opzione è abdicare e subire poi tutte

il cordoglio del Gruppo dell'Ulivo, ma credo possa dirsi il cordoglio del Senato, senza distinzione di Gruppi. Chi avrebbe moralmente più titolo a parlare è Rosa Villecco Calipari, ma ben comprendo le ragioni di umana commozione e ricordo che la inducono a rinunciarvi. Voglio dire anzitutto che né il Governo, né il Parlamento, ogni volta che si è trattato della missione internazionale in Afghanistan, hanno mai sottostimato la gravità, i rischi e le incognite della partecipazione italiana. Quella partecipazione risponde a finalità che non sono rinunciabili se l'Italia vuole contribuire, in modi proporzionati al suo ruolo internazionale, al processo di stabilizzazione in un'area che è cruciale per il futuro dell'Europa e del Pianeta. È del tutto evidente che la soluzione del caso afgano non sarà e non potrebbe essere militare, ma è altrettanto evidente che, sia la ricostruzione di quel disgraziato Paese, sia l'estirpazione delle basi del terrorismo internazionale, non sono possibili se l'organizzazione delle Nazioni Unite e, per suo mandato, l'Alleanza Atlantica, non sono nelle condizioni di stabilire i requisiti minimi della sicurezza. A ciò provvedono i militari del contingente italiano, cui non soltanto oggi nell'ora del lutto, ma ogni giorno, deve andare l'apprezzamento e il rispetto della nazione. L'Afghanistan è il banco di prova del multilateralismo ai fini della costruzione della pace e il maggior banco di prova per la nuova missione dell'Alleanza atlantica. Come ha ricordato poco fa il collega Selva, domani si apre in Islanda la sessione annuale dell'Alleanza,

devono valere (a suo tempo fu approvato un ordine del giorno in proposito qui nell'Aula del Senato) anche nelle procedure da adottare nei casi sempre più frequenti di sequestro: procedure concordate per proteggere i sequestrati dalle indiscrezioni e dalle fughe di notizie che possono aggravarne il pericolo - come purtroppo credo sia avvenuto in occasione del sequestro del 24 settembre - e per la collaborazione più efficace tra i contingenti della missione multinazionale e con il governo locale; infine, onorevole Sottosegretario, anche per fare luce sulle cause e sulla dinamica dei sequestri e del loro esito. passato in quest'Aula - lo ricordiamo tutti - si è discusso della preferibilità delle procedure da adottare per risolvere i sequestri: dalla trattativa, che diffonde ombre che poi sono difficili da dissipare e che richiede compensazioni di cui quelle finanziarie sono soltanto le più ammissibili, alla soluzione di forza, che comporta sempre un alto rischio per l'incolumità degli ostaggi. Nel caso del sequestro del 24 settembre, come abbiamo sentito dal rappresentante del Governo, la dinamica non lasciava altra scelta che la soluzione di forza.

ai modi della liberazione, all'origine cui va attribuito il ferimento degli ostaggi. Ripeto in questa sede la domanda che ho fatto al ministro Parisi in Commissione difesa perché credo, signor Presidente - me lo lasci dire - che quando un soldato muore in servizio nell'adempimento del proprio dovere, non solo la sua famiglia ma il popolo italiano ha diritto di conoscere tutta la verità. Siamo certi dalla sensibilità del Governo a questo proposito ed esprimiamo la nostra solidarietà alle Forze armate e al Servizio di informazione e sicurezza militare, un commosso augurio ai feriti e una profonda vicinanza alla famiglia del caduto; onore al maresciallo Lorenzo D'Auria, caduto al servizio militare nel nome della pace.

la morte di un servitore dello Stato, come veniva ricordato nel dibattito, che impone a tutti non solo una riflessione, ma anche una sottolineatura rispetto al lavoro che molti uomini e anche donne svolgono in aree difficili per cercare di rendere questo mondo un po' meno difficile di quanto in realtà sia e portare aiuto a chi vuole la pace e pensa di ricostruire il proprio Paese.

Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori, con riferimento all'apertura della sessione di bilancio che avverrà di qui a poco, poco, per fare presente all'Assemblea, e quindi testimoniare anche con la registrazione dell'intervento, una questione estremamente rilevante che attiene in particolare al decreto‑legge che costituisce parte della manovra finanziaria. Lo dico, Presidente, perché attiene proprio alle modalità

e in maniera molto determinata da parte della Corte costituzionale con una sentenza che risale al maggio di quest'anno, la n. 171 del 2007.

dire, funzionale e procedimentale tale da consentirle, ancorché non siano stati convertiti, di valutare i presupposti di necessità e urgenza così come previsto dall'articolo 77 della Costituzione,

ci sarà, ripeto, un dibattito in Commissione e in Aula), è anche necessario che gli emendamenti rispondano agli stessi canoni, perché il procedimento di approvazione dei decreti-legge è strutturato proprio sui presupposti che devono stare alla base di questo eccezionale conferimento al Governo Governo di un potere fondamentale: il potere legislativo. Voglio allora invitare la Presidenza, e tramite di essa la Presidenza della Commissione, a fare particolarmente attenzione alle questioni di ammissibilità, perché la sentenza della Corte ci richiama tutti a un dovere di rispetto dei canoni costituzionali. Non si possono utilizzare gli strumenti eccezionali previsti dalla Costituzione per eludere le norme ordinarie previste dalla Costituzione medesima. Questo è il succo della sentenza della Corte. Mi spiace che questo decreto-legge che il Governo ci ha consegnato, e che avrebbe potuto rappresentare un primo riconoscimento della sentenza della Corte, la disattenda invece, a mio avviso,

quello che viene definito l'ecomostro di Alimuri, uno scheletro in cemento armato costruito nel 1964 in un'area naturalistica di grande pregio ambientale nel Comune di Vico Equense, in provincia di Napoli, sulla costiera sorrentina: una concessione edilizia rilasciata nel 1964 e revocata nel 1971, rispetto alla quale c'è stata una serie di sentenze successive che non hanno mai riconosciuto la legittimità di questo

dell'immobile (quindi di un manufatto illegale in località Alimuri a Vico Equense) dispone l'abbattimento della struttura di 18.000 metri cubi ed il ripristino del fronte a mare e del costone alle spalle del manufatto. Fermo restando che gli interpellanti sono d'accordo che, dopo quarant'anni, si ponga fine e si abbatta quel manufatto, tuttavia vi sono diverse clausole all'interno di quell'accordo che appaiono, a nostro avviso, fortemente discutibili, perché eccessivamente vantaggiose per la società proprietaria dell'immobile. In primo luogo, la società, la SaAn, ha ottenuto che Stato e Regione finanzino per oltre la metà - 600.000 euro su un 1.100.000 euro complessivi - le spese di demolizione e consolidamento del costone; un'altra clausola include la possibilità che un qualsiasi aumento dei costi durante le operazioni di abbattimento vada a carico degli enti pubblici firmatari dell'accordo. È plausibile che lo Stato e la Regione si facciano carico di tali spese, tenuto conto che la lievitazione dei costi è molto probabile considerato che siamo in una zona ad altissimo rischio idrogeologico, la zona rossa della fascia costiera della della Provincia di Napoli? In secondo luogo, in base a quell'accordo la società, una volta demolito quel manufatto, ha diritto a una permuta in cubatura, ossia le viene data la possibilità di costruire, negli ambiti 4 e 5 del piano regolatore del Comune di Vico Equense, un nuovo albergo con le stesse cubature del manufatto illegale. Nell'accordo è scritto testualmente: "la delocalizzazione della volumetria equivalente a quella del manufatto da abbattere". Un primo dubbio riguarda il fatto che ci troviamo davanti ad uno scheletro non ad una struttura quindi non vi è già un albergo in funzione, e ci sono diverse sentenze del Consiglio di Stato che sanciscono che un rustico non completato non dà diritto a volumetria, a cubatura alcuna per i proprietari. metri cubi, pertanto, correttamente non sono inseriti nel piano regolatore del Comune di Vico Equense, quindi l'eventuale riconoscimento dell'accordo del 19 luglio consentirebbe la costruzione di nuovi 18.000 metri cubi su una zona, come la penisola sorrentina, che ha problemi serissimi di di natura opposta, di decongestionamento, di riduzione dei volumi, se si vuole rendere anche la sicurezza oltre che la vivibilità di quel territorio. Tra l'altro, c'è il rischio concreto che lo stesso nuovo albergo possa nascere in una zona vincolata, anche se ciò viene escluso nell'accordo, perché si dà facoltà ai proprietari dell'immobile da abbattere di individuare una area. La domanda sorge spontanea: nel caso in cui individuassero un'area e i proprietari non fossero disponibili alla vendita, in quel caso interverrebbe lo Stato con

non si comprende per quale motivo sia cambiata, a distanza di pochi mesi, la volontà di alcuni dei soggetti in campo, in particolare della Regione Campania che aveva, pochi mesi prima, nel mese di maggio,

considerando che nel 2004 la stessa società aveva scritto dimostrando disponibilità ad abbattere e al recupero solamente della metà dei volumi,

Signor Presidente, onorevoli senatori, il fabbricato individuato come "ecomostro" di Alimuri a ridosso della linea di battigia dell'omonima località, allo stato è un fatiscente scheletro in cemento armato costituito da due corpi multipiano contigui. Tale fabbricato è stato realizzato in virtù della concessione edilizia n. 67, rilasciata il 9 marzo 1964 dal Comune di Vico Equense. L'area di intervento è sottoposta a vincolo paesaggistico con decreto ministeriale del 5 novembre 1955, per cui l'allora Soprintendenza ai monumenti della Campania il 23 novembre 1963 ha rilasciato l'autorizzazione paesaggistica n. 5666. Già dall'inizio dei lavori le associazioni ambientaliste (in testa Italia Nostra) si sono attivate per impedirne la prosecuzione. L'11 giugno 1967 il Comune ha rinnovato la concessione edilizia n. 67 del 1964 e ha limitato la struttura a la struttura a «soli» 50 vani e accessori, stabilendo che l'altezza della stessa non dovesse superare i 16 metri. La nuova licenza edilizia n. 68 è stata rilasciata dal Comune il 31 agosto 1968. La Soprintendenza di Napoli, con l'ordinanza n. 5122 dell'8 aprile 1971, ha intimato alla società proprietaria la sospensione dei lavori per essere scaduta, rispetto ai termini di validità quinquennale, l'autorizzazione paesaggistica del 23 novembre 1963. Con ordinanza del sindaco di Vico Equense del 2 aprile 1971 è stata disposta la sospensione dei lavori e con la successiva ordinanza comunale n. 40 del 28 maggio 1971 è stata disposta la demolizione della opere fino allora realizzate. I proprietari hanno promosso ricorso gerarchico al Ministero della pubblica istruzione, allora competente per la materia, contro l'ordinanza della Soprintendenza; il ricorso è stato accolto dal Ministero con la II del 12 giugno 1972, che ha dichiarato nulla l'ordinanza della Soprintendenza. A seguito delle denunce dell'associazione Italia Nostra, i responsabili delle opere sono stati sottoposti a procedimento penale. Il pretore di Sorrento, con sentenza del 4 dicembre 1972, ha assolto gli imputati per non aver commesso il fatto. Nelle more del contenzioso amministrativo, i lavori sono proseguiti fino alla configurazione che attualmente presenta la struttura. Dopo nutrita corrispondenza tra Comune e Regione, con il decreto n. 3796 dell'11 novembre 1976, il Presidente della Giunta regionale ha annullato le licenze edilizie del 1964 e del 1968, poiché rilasciate in violazione dello strumento urbanistico allora vigente. A seguito di ricorso proposto dalla parte contro tale deliberazione, il TAR della Campania, con la sentenza n. 568 del 1979, ha dichiarato illegittimo il provvedimento regionale, perché emesso oltre i 18 mesi dal compimento dell'accertamento delle violazioni. Il 21 dicembre 1979 la Regione ha avanzato ricorso al Consiglio di Stato, che, con la sentenza n. 724 del 19 ottobre 1982, ha confermato il positivo giudizio del TAR. Con nota del 2 aprile 1986, l'allora società proprietaria ha comunicato la ripresa dei lavori*,* ma il Comune di Vico Equense, il 15 maggio 1986, ha diffidato la stessa dal riprendere le opere fino al consolidamento del retrostante costone confermato la sospensione dei lavori fino all'esecuzione di tale consolidamento, ad oggi non ancora realizzato. Inoltre, con l'ordinanza n. 26/86 del 12 maggio 1986, ancora vigente, ha vietato il transito e la sosta di persone o cose nell'area ove è posto il manufatto. L'Amministrazione comunale, con la delibera n. 27 dell'1 marzo 2001, ha espresso l'indirizzo di demolire lo scheletro in cemento armato in argomento, nel frattempo trasformatosi in una fatiscente struttura che, oltre a deturpare fortemente il paesaggio costiero, costiero, è diventata ritrovo per lo spaccio e l'uso di stupefacenti. Nel 2003*,* presso il settore politica del territorio della Regione Campania, è stato attivato un tavolo tecnico, con la presenza della Regione, dei Comuni di Vico Equense e di Meta e della società SaAn, per studiare la possibilità di demolire l'ecomostro con la realizzazione, in sostituzione, di strutture balneari di tipo stagionale e la delocalizzazione in altro sito del Comune di Vico Equense delle volumetrie da demolire. Il 16 novembre 2006, la Giunta comunale di Vico Equense, preso atto dell'avvio, da parte della Regione Campania, del tavolo tecnico finalizzato alla riqualificazione dell'area in località Conca di Alimuri, ha ratificato gli impegni afferenti al consolidamento del costone roccioso soprastante l'area e si è determinata, per la demolizione del manufatto esistente e, delocalizzazione dello stesso in altro sito del territorio comunale. L'11 maggio 2007, la Soprintendenza di Napoli e Provincia e l'Assessorato all'urbanistica della regione Campania hanno avviato il procedimento per l'eventuale esercizio dei poteri *ex* articolo 21 *quinquies* della legge n. 241 del 1990 di revoca degli atti autorizzativi precedentemente adottati afferenti alla realizzazione del manufatto in argomento. La società proprietaria del manufatto si è resa disponibile ad assumere gli oneri economici connessi alla demolizione del manufatto, così come alla riqualificazione dell'area, mentre il Comune di Vico ha comunicato che l'Amministrazione provinciale, competente per la materia, con delibera del 3 agosto 2006 aveva approvato il progetto generale di consolidamento del costone di Alimuri, per l'importo complessivo di 5 milioni di euro. Con l'accordo firmato il 19 luglio 2007 tra il Ministro per i beni e le attività culturali, il Presidente della Giunta regionale della Campania, il Presidente dell'Amministrazione provinciale di Napoli e il Sindaco del Comune di Vico Equense si è stabilito, tra l'altro, che la spesa per il consolidamento del tratto di costone necessario per poter effettuare in sicurezza le operazioni di demolizione dell'ecomostro è stata quantificata in circa 800.000 euro. Tale consolidamento rientra tra le competenze istituzionali della Regione e, per delega di questa, della Provincia. Lo stesso costone, tra l'altro, non è proprietà della società SaAn. L'accordo del 19 luglio 2007 prevede che il relativo onere economico sia a carico della società proprietaria dell'ecomostro per 500.000 euro e a carico dell'Amministrazione regionale per 300.000 euro. Il Ministero per i beni e le attività culturali si è fatto carico dell'abbattimento dell'ecomostro e lo sgombero delle relative macerie, operazione quantificata in 300.000 euro e rientrante tra le competenze istituzionali del Ministero. Questo accordo comporta che la società proprietaria dell'ecomostro si farà carico di una cifra maggiore di 200.000 euro rispetto a quanto le spetterebbe per la demolizione e lo sgombero delle macerie, cifra che, ovviamente, va detratta dagli impegni economici a carico della pubblica amministrazione. Gli eventuali maggiori costi del consolidamento del costone sono legati esclusivamente all'estensione dell'area di consolidamento da realizzare. Solo nel caso in cui si prevedesse di consolidare una superficie di costone maggiore di quella necessaria alle operazioni di abbattimento, gli oneri connessi sarebbero, per competenza, a carico dell'Amministrazione regionale. È opportuno chiarire che l'ammissibilità della edificazione di una nuova struttura edilizia in compensazione di quella da demolire discende dalla legittimità della costruzione esistente. Del resto, già il tavolo tecnico attivato dal settore politica del territorio della Regione Campania nel 2003 ha assunto tra gli obiettivi la delocalizzazione della volumetria da demolire in altro sito del Comune di Vico Equense. Per quanto concerne l'area di sedime della struttura da demolire, va segnalato che l'accordo del 19 luglio 2007 non prevede la realizzazione di alcuna struttura ricettiva, ma di strutture ricreative stagionali (per la balneazione) di facile rimozione e di bassissimo impatto ambientale (servizi igienici e spogliatoi, per esempio). Assicuro l'onorevole senatore interrogante che il Ministero ha comunque avviato ulteriori verifiche giuridico-amministrative per accertare se vi siano percorsi tecnico-procedurali che risultino più vantaggiosi per lo Stato e gli enti interessati e consentano di migliorare ulteriormente lo scenario che ho appena delineato. È uno scrupolo in più e daremo volentieri informazione al Parlamento in ordine a questi ulteriori approfondimenti che stiamo operando. Infine, l'area dove andrebbe edificata la volumetria da demolire, ricadendo nel territorio comunale di Vico Equense, è sottoposta a vincolo paesaggistico. La nuova localizzazione non è contemplata nell'accordo del 19 luglio 2007. Ovviamente la stessa va attentamente valutata per l'elevato valore paesaggistico del territorio comunale di Vico Equense. A tale scopo il Ministero per i beni e le attività culturali si è fatto carico di impegnare le Amministrazioni firmatarie dell'atto alla costituzione di un tavolo tecnico finalizzato a valutare la proposta relativa alla delocalizzazione della volumetria da demolire, che potrà essere ricostruita esclusivamente nelle zone territoriali 4 o 5 del vigente piano urbanistico territoriale della penisola sorrentino-amalfitana, zone nelle quali lo stesso piano prevede la possibilità della creazione di nuove volumetrie turistico-ricettive. Il tavolo tecnico è stato insediato il 24 luglio 2007 presso il Comune di Vico Equense e vede presenti, oltre alle Amministrazioni regionale e provinciale, anche il Ministero attraverso la direzione generale per i beni architettonici e il paesaggio, la direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Campania e la Soprintendenza di Napoli e Provincia.

anche perché nella sua ricostruzione, in larga parte riprendendo ciò che è scritto nell'interpellanza e anche quello che avevo esposto nell'illustrazione in modo abbastanza puntuale, c'è

non hanno attestato la legittimità delle licenze ma hanno semplicemente dichiarato che i termini entro cui si erano prodotti i ricorsi erano scaduti. Quindi, l'illegittimità dell'atto era del tutto palese. Del resto, uno scheletro che è rimasto in piedi per 43 anni il Governo potrebbe sollevare l'obiezione che forse la strada dell'azione giudiziaria o dell'atto di imperio per arrivare all'abbattimento avrebbe richiesto ancora qualche mese o qualche anno.

non l'ho detto in premessa ma sussiste anche un motivo di opportunità. Credo non sfuggirà al Governo che la proprietà dell'albergo ha

Signor Presidente, in merito alla questione delineata nell'atto parlamentare in esame, il Ministero della salute ha acquisito le necessarie informazioni dalle aziende ospedaliere interessate e dalla Federazione nazionale dei medici chirurghi e odontoiatri. Il complesso ospedaliero "San Giovanni-Addolorata" di Roma ha comunicato che al dottor Huscher è stato conferito l'incarico quinquennale di dirigente medico di secondo livello presso l'unità operativa diagnostica di chirurgia generale, a seguito di selezione effettuata da una commissione di esperti ai sensi dell'articolo 15-*ter* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Il sanitario è stato assunto in servizio in data 1° giugno 1998. Con delibera del 4 aprile 2004 il contratto è stato rinnovato per il periodo 1° giugno 2003-31 maggio 2008; successivamente, con deliberazioni del direttore generale del 4 e 26 marzo 2005, il contratto di lavoro è stato risolto per giusta causa, con effetto dal 16 maggio 2005. Tale risoluzione è intervenuta poiché al sanitario, in data 10 maggio 2004, sono stati notificati atti di citazione per errate cure, con la quantificazione del corrispondente risarcimento. L'azienda citata, inoltre, in data 3 novembre 2005, è venuta a conoscenza di cinque procedimenti penali a carico del dottor Huscher per i reati previsti dagli articoli 582, 583, 584 e 589 del codice penale, dei quali il professionista non aveva dato la debita informazione in occasione delle procedure per la selezione. L'azienda si è costituita in giudizio. Si segnala che in data 28 settembre 2007 la sezione lavoro del tribunale di Roma ha disposto con sentenza di reintegro la riammissione in servizio del citato professionista. Relativamente al servizio prestato a Milano presso l'azienda ospedaliera «Ospedale San Carlo Borromeo», era stato conferito un incarico biennale a tempo determinato, sulla base del *curriculum vitae* e dell'esperienza professionale dell'interessato; peraltro, il medico suddetto ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico dal 1° febbraio 2007. Il direttore generale dell'azienda sanitaria locale n. 3 "Centro Molise" di Campobasso ha precisato che relativamente ai presunti impatti chirurgici «altamente demolitivi», gli stessi, gli stessi, potendo essere compatibili solo con situazioni cliniche «particolarmente critiche», costituiscono, nell'autonoma valutazione del paziente che intende sottoporsi ad intervento, un rischio ampiamente calcolato, alla luce anche del cosiddetto consenso informato, obbligatorio per legge. In tema di tasso di mortalità, lo stesso direttore ha inteso rilevare il rapporto direttamente proporzionale tra la criticità chirurgica e il relativo intervento; ha sottolineato inoltre che, per quanto riguarda le ipotesi di reato, è d'obbligo il massimo rispetto «tanto per il lavoro degli inquirenti, quanto per la salvaguardia dell'immagine del professionista». Per quanto concerne la determinazione di assegnare al citato professionista l'incarico presso il Presidio ospedaliero «Ferdinando Veneziale» di Isernia, il direttore generale ha precisato che, dopo aver verificato la disponibilità dello stesso a prestare la propria attività nel Molise, ha inteso cogliere tale opportunità al fine di assicurare ai cittadini molisani, «nella malaugurata ipotesi in cui ne dovessero avere necessità, un'opportunità in più, non fuori o all'estero, ma in Molise e ad Isernia», anche al fine di incidere, consistentemente, sulla bilancia della mobilità sanitaria molisana, come nei fatti si sta verificando (secondo quanto affermato dallo stesso direttore sanitario), «in quanto la riduzione dell'emigrazione e l'aumento dell'immigrazione sanitaria stanno determinando un saldo attivo, mai come in questo momento non solo utile, ma oggettivamente necessario, alle finanze regionali». L'incarico al dottor Huscher di direttore dell'unità operativa di chirurgia generale presso il presidio ospedaliero citato è stato disposto, secondo l'azienda, «per chiara fama», avvalendosi degli strumenti previsti dalla normativa vigente, e trova fondamento nel rispetto dei princìpi inerenti all'affidamento di incarichi e nella necessità di garantire una professionalità non immediatamente acquisibile tramite le procedure concorsuali. La Federazione nazionale ordini medici chirurghi e odontoiatri ha comunicato che nei riguardi del sanitario, iscritto all'Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri di Brescia dal 20 febbraio 1976, lo stesso Ordine provinciale ha disposto un procedimento disciplinare per i reati di cui agli articoli 582, 583, 584 e 589 del codice penale;

sono in parte soddisfatto per le notizie apprese stasera, ma il problema è molto più grave di quello che appare. appare. Il professionista in oggetto ha ricevuto oltre 64 avvisi di garanzia. Il tasso di mortalità nell'ospedale di Isernia, dove è stato nominato, è notevolmente aumentato. L'elemento di bilancio della mobilità sanitaria non si è ridotto, si è ridotto per i molisani della Provincia di Isernia che vanno altrove,

Il motivo di tutto questo è legato non solo agli interessi del dottor Huscher; si utilizza la chiara fama quando in realtà la legge è molto esplicita riguardo alla nomina dei primari di responsabilità di unità operative complesse e, nel caso specifico, non vi è stato

appunto nell'ospedale di Isernia senza avere alcun rapporto con quell'ospedale, utilizzando un contratto su interventi di 500.000 euro che il dottor Huscher dovrebbe effettuare per attivare un progetto per l'applicazione della chirurgia laparoscopica che dovrebbe essere utilizzata all'interno di quella struttura. Ciò che sta accadendo in quell'ospedale ormai grida vendetta sul piano della serietà e della correttezza degli interventi.

Il Molise è la seconda Regione sul piano dei costi complessivi che presenta un disavanzo sanitario enorme. Come è possibile pensare che mentre è in vigore il blocco delle assunzioni per il piano

Ebbene, tutto questo sta accadendo e da parte del Ministero della sanità ci vorrebbe un controllo maggiore in questa particolare direzione. Nonostante la presenza del rappresentante del Ministero della sanità e di quello del Ministero del del Ministero del tesoro, abbiamo una situazione complessiva ancora più drammatica di quella precedente. Non vi sono piani di rientro che, comunque, non vengono rispettati. Vi è una situazione difficile, che la popolazione della Provincia di Isernia continua a pagare per il senso di responsabilità di un presidente che assume solo parenti, affidando anche incarichi per unità complesse, ma che si è contornato di un comitato d'affari che sulla sanità,

per la salute*. Preliminarmente si ribadisce l'impegno del Ministero nella lotta a tutte le possibili forme di contraffazione che possono costituire un danno alla salute dei cittadini, come si è avuto occasione di precisare nelle risposte ad altri atti parlamentari. Relativamente al problema farmaci, in Italia il controllo sulla produzione si svolge con regolarità e copre anche gli aspetti critici che hanno causato in altre Nazioni i decessi citati dal senatore Gramazio. La normativa europea, ai sensi della direttiva 2001/CE/83, recepita nel nostro Paese con il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, prevede per i titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci l'obbligo di controlli e verifiche stringenti, realizzati attraverso l'applicazione corretta delle norme di buona fabbricazione dei medicinali, che vengono a loro volta monitorate avvalendosi delle ispezioni effettuate dall'Agenzia alle quali sono soggetti i produttori di farmaci e di materie prime farmacologicamente attive. L'Italia fin dal 1991 svolge regolari ispezioni presso i produttori. Nella lotta ai farmaci contraffatti, l'Italia è certamente all'avanguardia in Europa, avendo da tempo avviato una attiva cooperazione con l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e il Consiglio d'Europa (i due enti che più si occupano del tema a livello internazionale). L'AIFA ha anche individuato un coordinatore delle attività anticontraffazione, che segue, con la cooperazione dei Carabinieri NAS, i casi di interesse per l'Italia attraverso il collegamento con i punti di contatto internazionali. Tra le attività nazionali già in corso sul tema, coordinate dall'AIFA, ce n'è una particolarmente significativa, che riguarda il commercio illegale dei medicinali su Internet, che è una delle principali fonti di provenienza

La vigente normativa prevede la presenza di un bollino ottico su tutti i farmaci e la tracciatura dell'intera vita di un farmaco: la produzione, l'immissione in commercio, l'importazione, l'esportazione, la distribuzione e la vendita al pubblico sono subordinate ad un processo di autorizzazione o notifica e di vigilanza da parte del Ministero della salute, dell'Agenzia italiana del farmaco e delle Regioni e/o Province autonome e delle autorità da loro delegate. I farmaci presenti sul territorio nazionale sono dotati di un bollino ottico dell'Istituto poligrafico dello Stato e, pertanto, un'eventuale contraffazione implicherebbe anche la contraffazione di tale bollino. L'intero *iter* dei farmaci è stato delineato grazie al progetto sulla tracciabilità del farmaco, avviato con il decreto ministeriale 15 luglio 2004; tutti i soggetti autorizzati all'acquisto o alla cessione di un farmaco devono registrare tali operazioni e comunicarle alla banca dati sulla tracciabilità gestita da questo Ministero e dall'AIFA. Si ribadisce che proprio una possibile mancata quadratura dei flussi informativi fornisce preziose indicazioni, per le verifiche sul territorio, ai NAS che hanno accesso al progetto. La lotta alla contraffazione attualmente è mirata all'identificazione dei siti illegali in Italia ed all'estero che producono, distribuiscono o vendono anche via Internet farmaci contraffatti ad ignari cittadini e, talvolta, ad altrettante ignare organizzazioni umanitarie, ad una modifica delle norme vigenti con l'introduzione di nuove norme e sanzioni ed all'elaborazione di efficaci interventi di comunicazione sul rischio correlato all'acquisto di farmaci contraffatti. In tale ottica questo Ministero collabora sia con le altre amministrazioni nazionali coinvolte in tale lotta, quali l'AIFA, l'Istituto superiore di sanità, Comuni, sia con gli organismi internazionali. Il Ministero, inoltre, è rappresentato ai due tavoli tecnici di lavoro che hanno entrambi come obiettivo la lotta alla contraffazione e l'integrazione delle correlate attività. Il tavolo permanente delle istituzioni presso l'Alto commissariato per la lotta alla contraffazione intende acquisire, tramite il superamento della dispersione delle competenze, l'approfondimento della conoscenza del fenomeno complessivo della contraffazione, la messa a punto di una strategia di lotta e l'elaborazione di norme di carattere generale. Il tavolo tecnico istituito con la determinazione AIFA del 16 aprile 2006 ha come obiettivi prioritari l'approfondimento del fenomeno della contraffazione dei farmaci, la definizione di procedure analitiche per l'identificazione dei farmaci contraffatti, lo studio sui farmaci distribuiti via Internet, l'elaborazione di norme specifiche. Tale tavolo dovrebbe configurarsi come punto di riferimento per le segnalazioni dei casi di contraffazione e come referente italiano nel progetto "Impact" dell'OMS, relativo alla istituzione di una *task force* internazionale Si ritiene opportuno riferire, secondo quanto comunicato dal comando generale della Guardia di finanza, che i competenti reparti stanno vigilando con particolare attenzione sulle importazioni di merci provenienti dal Sud-Est asiatico, per gli elevati indici di rischio connessi all'introduzione nel territorio di merce contraffatta ovvero di contrabbando. L'attività operativa svolta al riguardo nel periodo gennaio 2006-maggio 2007 ha consentito di individuare illecite introduzioni di farmaci e medicinali provenienti dalla Cina costituiti da: 22.308 confezioni di medicinali; 4 chilogrammi di medicinali; 14.899 *blister* di capsule; 668 bustine di polvere granulato; 843 confezioni di creme; 250 confezioni di olio medicale; 135 confezioni di unguento medicale; 117 cerotti medicali; 159 confezioni di amuxicillina; 2.174 integratori; 330 fiale; 14 flaconi di collirio e 29 flaconi di medicine. Sono stati denunciati all'autorità giudiziaria 36 soggetti di origine asiatica per i reati, tra gli altri, di contrabbando aggravato, frode in commercio, commercio di medicinali guasti. In relazione all'interrogazione parlamentare, è stata segnalata la rilevanza di un'indagine di polizia giudiziaria sviluppata d'iniziativa dei reparti del comando provinciale di Catania nell'ottobre 2006. L'indagine ha tratto origine dalle investigazioni effettuate a seguito del sequestro di merce contraffatta presso un locale emporio di prodotti cinesi, che hanno consentito di rinvenire un vasto campionario di balsami, oli medicamentosi e lozioni. Le analisi svolte dall'Istituto superiore di sanità hanno evidenziato che i suddetti prodotti, da ritenere farmaci a tutti gli effetti, sono da considerarsi pericolosi per la salute, poiché tossici ed irritanti. L'autorità giudiziaria di Catania ne ha disposto il sequestro su tutto il territorio nazionale e sono stati denunciati 313 soggetti di nazionalità asiatica (di cui uno tratto in arresto) e sequestrate 49.000 confezioni di prodotti medicinali di origine cinese. Il comando citato ha ribadito che, tenuto conto delle pericolose conseguenze per la salute e la sicurezza dei consumatori derivanti da ulteriori possibili traffici illeciti, sono stati sensibilizzati i reparti del Corpo affinché venga adottata ogni possibile misura di presidio e salvaguardia del settore.

di migliaia di pezzi, ma anche ad uno sciroppo che, fabbricato in Cina, arriva in Sud America, viene rietichettato e riportato poi in Europa;

La risposta è stata alquanto fastidiosa, perché ha detto di avere solo 194 dipendenti e quindi di non avere le strutture delle uguali aziende che operano in altre parti d'Europa.

di prodotti medicinali che costano dal 50 al 60 per cento in meno. Si registra pertanto la situazione di mercato che ho voluto evidenziare. Mi permetterei altresì di fa rilevare ancora al nostro gentile Sottosegretario che nell'ultimo anno si è quintuplicato

richiamerei affinché la struttura preposta - cioè appunto l'AIFA - avesse un occhio di riguardo per Internet e denunciasse subito alla Guardia di finanza e ai NAS dei carabinieri la vendita di questi farmaci, che sono illegali perché non sono passati attraverso nessuno dei controlli

Con riferimento alla problematica rappresentata nell'atto parlamentare, si precisa preliminarmente che la sclerosi laterale amiotrofica è ricompresa nell'elenco delle malattie rare previste dal decreto ministeriale del 18 maggio 2001, n. 279, e successive modifiche. I soggetti affetti da tale patologia hanno diritto, in regime di esenzione, alle prestazioni necessarie, secondo criteri di appropriatezza ed efficacia, per il trattamento e il monitoraggio della malattia rara accertata e per la prevenzione di ulteriori aggravamenti, fatta salva la facoltà per le autorità regionali di stabilire provvidenze aggiuntive a favore di tali ammalati. Fin dall'inizio del suo mandato governativo, il Ministro della salute ha avuto una particolare attenzione per questa categoria di pazienti. Si segnalano pertanto le recenti iniziative adottate al riguardo. In data 1° agosto, la Conferenza Stato-Regioni ha ratificato in via definitiva il provvedimento con il quale il Ministro della salute ha destinato 10 milioni di euro, ripartiti tra le Regioni, per l'acquisto di comunicatori vocali (sistemi di comunicazione aumentativa alternativa) a favore dei pazienti affetti da SLA o da altre gravi patologie croniche ad andamento degenerativo, che comportino la perdita della parola, lasciando intatte, peraltro, le capacità cognitive. Nelle fasi più avanzate della malattia, quando solamente i movimenti oculari riescono a creare un rapporto tra i pazienti e il mondo circostante, la tecnologia può fare molto per aiutarli ad intensificare questo rapporto; i dispositivi a controllo oculare garantiscono tutto ciò grazie ad una telecamera connessa ad un *computer* e ad un *software*, consentendo di scrivere, navigare in Internet, leggere, scrivere e spedire *e-mail*, comandare luci e apparecchi domestici. Il ministro Livia Turco ha voluto dare una risposta concreta a una domanda pressante proveniente dalle associazioni di tutela più impegnate nella lotta a questa patologia, a sostegno della qualità della vita anche nelle fasi più dolorose. Inoltre, si precisa che tra pochi giorni entrerà in vigore il decreto, in data 2 agosto

concernente la semplificazione degli adempimenti amministrativi per le persone con disabilità, individua l'elenco delle patologie escluse dalle visite di controllo per la verifica della permanenza dello stato di invalidità, qualora sia stato già riconosciuto il diritto alla indennità di accompagnamento o di comunicazione. Il decreto include dodici voci, relative a condizioni patologiche che determinano una grave compromissione dell'autonomia personale e gravi limitazioni alla vita comunitaria. Per tali patologie non saranno più necessari esami di controllo e di verifica per la continuità del riconoscimento dello stato invalidante, sulla base di due elementi: la gravità della condizione e l'impossibilità del miglioramento, in base alle attuali conoscenze mediche. Le dodici voci individuate da un gruppo di esperti del Ministero della salute, dell'INPS e delle organizzazioni di tutela dei disabili, componenti della commissione ministeriale «Salute e disabilità», includono tra l'altro patologie come quelle del rene in trattamento dialitico non trapiantabile, le patologie oncologiche con compromissione secondaria di organi e apparati, le patologie del fegato non trapiantabili, i *deficit* totali della visione e dell'udito, congenito o insorto nella prima infanzia. La relativa documentazione sanitaria indicata nel decreto suddetto andrà richiesta alle commissioni che si sono espresse in favore delle indennità citate o agli interessati, qualora non sia stata acquisita da parte delle commissioni. Infine, per garantire la massima aderenza ai bisogni dei cittadini e allo sviluppo delle conoscenze e delle nuove acquisizioni scientifiche e tecnologiche, il decreto prevede che l'elenco delle patologie, per le quali non è più necessario ripetere visite di controllo o di revisione, venga verificato con cadenza annuale. Con riferimento alla richiesta, contenuta nella interrogazione, di includere i soggetti affetti da LIS (*Locked-in delle attività della commissione ministeriale SLA, estendendone gli eventuali benefici, (percorsi diagnostico-terapeutico-assistenziali, piani terapeutici, linee guida per la presa in carico, assistenza a domicilio), si precisa che la stessa commissione ministeriale ha adottato come criterio guida dei propri lavori non solo la diagnosi di partenza ma anche la perdita di funzioni, in linea con le indicazioni più accreditate in letteratura scientifica. Tale criterio, che ha consentito di includere i pazienti suddetti, suddetti, è stato già utilizzato per l'Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in materia di obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per l'attuazione del Piano sanitario nazionale 2006-2008, sancito in data 1° agosto 2007 in sede di Conferenza Stato-Regioni, concernente la linea progettuale relativa alla «Facilitazione della comunicazione nei pazienti con gravi patologie neuromotorie» con la quale è stata vincolata, come sopra precisato, una quota di 10 di 10 milioni di euro, da ripartirsi tra le Regioni per l'acquisto di sistemi di comunicazione aumentativa alternativa. Si sottolinea al riguardo che il progetto è rivolto ad un primo *target* di pazienti, tra quelli con fonazione di grado 2 (sostanziale perdita della parola) e motilità di grado 4 (tetraparesi): l'intervento prevede espressamente tra i destinatari anche «i «i pazienti con sindromi *post* traumatiche per lesioni cervicali alte che esitano in tetraparesi completa con dipendenza dal ventilatore meccanico e quelli con sindrome Locked-in». In analogia, sono stati adottati criteri inclusivi dei pazienti con LIS anche per quanto attiene il già citato decreto interministeriale del 2 agosto 2007. Per quanto riguarda la possibilità di estendere a tutto il territorio nazionale le provvidenze che alcune Regioni riconoscono per l'assistenza ai malati di SLA, la suddetta commissione ha ricevuto dal Ministro della salute il mandato di elaborare linee guida per la presa in carico dei pazienti SLA, da sottoporre in seguito alle necessarie valutazioni delle Regioni, nelle sedi istituzionali opportune, allo scopo di verificarne la possibile adozione su tutto il territorio nazionale. Più specificamente, per quanto concerne la revisione del piano assistenziale del signor Steccato, come richiesto nell'atto parlamentare, si precisa che su questa particolare vicenda è stata richiamata l'attenzione dell'assessorato per le politiche della salute della Regione Emilia-Romagna. Il Ministero ha ricevuto a questo proposito una comunicazione del direttore sanitario della ASL di Piacenza che, per quanto attiene l'assistenza domiciliare, sostiene che la permanenza a domicilio per la quale ha optato il signor Steccato si è resa possibile garantendo a totale carico dell'azienda USL e del Comune il massimo di qualità e sicurezza assistenziale attraverso: l'installazione di un montascale; l'adeguamento della camera da letto a locale di assistenza sanitaria attraverso la fornitura di un letto elettrico, di un sollevapazienti sollevapazienti a muro e a carrello, di ossigeno liquido, di aspiratore, di saturimetro, di pompa nutrizionale enterale... ...la fornitura di una carrozzina elettrica e di tutti gli ausili per la movimentazione e il posizionamento del paziente; la fornitura di tutti i farmaci e presidi sanitari necessari; l'erogazione di prestazioni assistenziali consistenti in ADI di terzo livello, con rivalutazione trimestrale e accesso del medico di medicina generale due-tre volte la settimana; accessi infermieristici concordati direttamente con il medico di medicina generale e la famiglia e in ogni caso su chiamata per bisogni improvvisi;

per tre ore per sei giorni la settimana e per 1,5 ore per i giorni festivi; disponibilità di consulenze medico-specialistiche programmate e urgenti; dispositivo di chiamata automatica al «118» per situazioni di urgenza. Il signor Steccato beneficia dell'assegno di cura di 23 euro giornalieri, importo massimo fissato dalla per disabili gravissimi in trattamento domiciliare, oltre all'assegno di accompagnamento ai sensi della legge n. Su richiesta della moglie del signor Steccato di una integrazione temporanea all'assistenza che attualmente viene fornita, dovendo la signora sottoporsi ad un intervento chirurgico con conseguente periodo di convalescenza, è stata concordata con la signora la seguente modalità assistenziale: l'Azienda USL e il Comune di Piacenza si faranno carico di concedere un contributo assistenziale straordinario di € 880 euro mensili per tre mesi, eventualmente prorogabile qualora venga valutata non conclusa la fase di convalescenza della signora. Tale contributo, necessario per sostenere l'acquisizione di un assistente familiare che possa non solo aiutare e affiancare la signora nell'assistenza al marito, ma anche, sulla base delle indicazioni ricevute, gestire le manovre assistenziali di base necessarie, sarà erogato dal Comune di Piacenza a fronte della presentazione da parte della signora Ricetti della documentazione relativa alla regolarità contrattuale dell'assistente famigliare e alla spesa sostenuta.

che riguarda un uomo, Gian Piero Steccato, che - purtroppo per lui - è lucido e ha ascoltato quello che ha detto il rappresentante del Governo: comunica solo con un polpastrello e quindi non ha la possibilità di indignarsi, come potrebbe fare chiunque tra noi conoscesse il suo caso. Nel gioco delle parti parlamentari di solito è normale che l'opposizione esprima insoddisfazione per le risposte fornite dal Governo. È difficile esprimere indignazione in un'Aula deserta,

di chiamare i funzionari per dire loro «Queste cose non me le fate dire più, perché ci vuole un po' di umanità e non solo di burocrazia», perché qui si tratta di parlare della vita delle persone. Non è vero quello che ci ha raccontato, altrimenti altrimenti potremmo anche fare un altro gioco, se non parlassimo di una vicenda tragica. La inviterei a ripetere con parole sue quello che ha detto, perché queste vicende vanno vissute. Lei ci ha raccontato delle cose che probabilmente ha in animo di far succedere: nessuno ci ha spiegato come accadranno, se la situazione resterà quella che abbiamo denunciato. Presidente, mi consenta una annotazione. A me dispiace che sulla questione non sia venuta qui a rispondere in prima persona il Ministro della salute. Ho avuto la ventura, forse non per il Paese, di occupare quel posto prima del ministro Turco e credo che si potrebbe chiedere una rapida testimonianza a tanti malati di questo Paese, se il Ministro in persona non si occupasse di queste questioni. Cito il caso Crisafulli di Catania, il più famoso, ma potrei citare tantissimi altri casi di malati gravissimi che avevano il diritto di sapere che le istituzioni li consideravano persone vive,

e non vuole morire - e la risposta è quella, burocratica, che ci ha portato qui il signor Sottosegretario. Ci ha parlato a lungo della sindrome della sclerosi laterale amiotrofica, che è cosa diversa da quella di cui stiamo parlando.

a comunicare con un polpastrello. Ve ne sono cinque o sei casi nel nostro Paese, un centinaio in tutto il Pianeta: ci si viene a dire che è stata istituita la Commissione per la sclerosi laterale amiotrofica (che è un dovere, ed ha fatto bene, in questo caso, il Ministero ad istituirla), ma vorrei ricordare che quei 10 milioni di euro prevedono progetti personalizzati per quel tipo di sindrome e non ancora per questo. Le carte, da questo punto di vista, sono chiare. Vede, signor Sottosegretario, i comunicatori vocali, cui lei ha fatto riferimento, non sono disponibili per Gian Piero Steccato: questa è la prima bugia che le hanno fatto dire. In secondo le hanno fatto dire un'altra cosa, ma non ho dubbi che ciò non sia dipeso dalla sua volontà, perché lei fa il suo mestiere, viene qui, legge delle carte e poi se le riporta. Chieda ai funzionari del Ministero che le hanno preparato queste carte, la prossima volta, di approfondire quello che dicono. Qui viene rinfacciata ad un malato gravissimo la somministrazione dei farmaci: deve ringraziare, il signor Steccato? Deve ringraziare che il servizio universale garantisce in questo Paese i farmaci a chi è malato? La realtà, vuole sapere com'è? I farmaci vengono forniti una volta al mese e spesso mancano i prodotti specifici o urgenti

Ma davvero stiamo scherzando? Allora, signor Presidente, capisco che abbiamo limiti di tempo e non voglio assolutamente violarli, perché i Regolamenti sono quelli che sono. Ho intenzione, sulla questione, di continuare a tenere alto il livello di attenzione delle istituzioni: spero di riuscirci. Vorrei capire se anche il Presidente della Repubblica, che si sperticò in messaggi pubblici nei confronti di Welby e del suo diritto a morire, vorrà fare la stessa cosa che ho fatto io. Sono andato, a nome del mio movimento politico, a incontrare la sofferenza: sono andato a Piacenza. Vada il Sottosegretario, accompagni il suo Ministro, si faccia accompagnare dal Direttore della ASL della Regione amica, accompagni il Presidente della Repubblica ad incontrare questo malato: veda che cosa accade ad una persona che si trova abbandonata e vorrebbe semplicemente trovare nelle istituzioni una parola di conforto che dimostri quanto queste gli sono vicine per il suo diritto di vivere. Vergogna per questo Governo!

com'è noto al senatore interrogante, l'articolo 11, comma 9, della legge n. 124 del 1999 ha ricondotto ad ordinamento, a decorrere dall'anno scolastico 1999-2000, i corsi a indirizzo musicale, autorizzati in via sperimentale nella scuola media e funzionanti nell'anno scolastico 1998-1999. Con decreto ministeriale del 6 agosto 1999, n. 201, sono state stabilite le tipologie di strumenti musicali insegnati, i programmi, gli orali, le prove d'esame, l'articolazione delle cattedre ed è stata istituita l'apposita classe di concorso. Il succitato decreto ministeriale è tuttora vigente e sarà oggetto di un'attenta valutazione in occasione della nuova definizione delle classi di concorso, che verrà operata nell'ambito della loro revisione, in coerenza con il nuovo quadro ordinamentale di riferimento. È altresì noto all'onorevole interrogante che, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo d'istruzione, sono state recentemente diramate alle scuole indicazioni per il *curriculum*, che saranno oggetto di sperimentazione fino all'anno scolastico 2008-2009. Nei due anni di sperimentazione, le indicazioni costituiscono il quadro culturale di riferimento e non comportano modifiche di carattere ordinamentale, che si attueranno solo al termine della sperimentazione. In occasione della revisione degli assetti ordinamentali, che sarà effettuata, come già riferito, al termine della sperimentazione, sulla base delle risultanze che da esse emergeranno, la richiesta avanzata dall'onorevole interrogante sarà tenuta nella debita considerazione. In tal senso peraltro è la risposta, alla quale si fa riferimento nell'interrogazione parlamentare in discussione, fornita in data 15 dicembre 2006 all'Unione nazionale arte musica spettacolo.

Pascarella, però devo fare qualche riflessione che mi porta a non potermi dichiarare pienamente soddisfatto. Do comunque atto al Sottosegretario d'avere inquadrato molto bene il problema. La mia riflessione va in tre direzioni. Il mandolino fu escluso dall'insegnamento nelle scuole medie dall'elenco allegato al citato decreto ministeriale

rispetto al fatto che magari qualcuno sostiene - io non sono d'accordo - che si trattava di un insegnamento poco richiesto o poco praticato? In secondo luogo chiedo di verificare se è

con uno sforzo del gruppo di lavoro appositamente insediato per il riordino complessivo delle classi di concorso, vi è la possibilità di inserire il mandolino in quei programmi, in quelle classi di concorso sin dal prossimo anno scolastico 2008-2009. Credo che faremmo un buon servizio all'integrazione interdisciplinare e all'arricchimento dell'insegnamento obbligatorio dell'educazione musicale. Infine, l'insegnamento del mandolino è stato chiesto da migliaia di utenti, anche perché ha grande valore storico e culturale non più soltanto in alcune aree del Paese come Napoli e Cremona, che hanno un'importante realtà artigianale nel campo della liuteria con un grande valore economico. Il fatto stesso che vi sono oggi quattro conservatori in Italia Napoli, Bari, L'Aquila e Padova - che insegnano il mandolino è segno di una crescente importanza di questo strumento. Quindi concludo

con direttiva del 28 luglio 2005, n. 68, sono state fornite indicazioni ai competenti direttori generali degli uffici scolastici regionali per l'indizione e la gestione delle gare finalizzate alla stipula di "contratti normativi" con i quali regolamentare, nell'ambito delle risorse appostate nei bilanci dei singoli uffici scolastici regionali,

delineare un percorso omogeneo, finalizzato a favorire l'adozione, da parte dei singoli uffici scolastici regionali, nell'ambito dei quali sono svolte le attività esternalizzate, di comportamenti univoci e condivisi, è stata allegata alla direttiva la documentazione di gara predisposta in collaborazione con il Ministero dell'economia e delle finanze. Il competente ufficio scolastico regionale della Toscana ha precisato di aver proceduto all'indizione della gara regionale per l'affidamento del servizio di pulizie ed altre attività ausiliare con bando pubblicato in data 23 maggio 2007, secondo le disposizioni contenute nella direttiva n. 68 del 28 luglio 2005, sia per quanto riguarda le attività ed i servizi da erogare, sia per quanto riguarda il mantenimento dei livelli di esternalizzazione dei servizi stessi. Il medesimo ha affermato che non corrisponde a realtà che l'ufficio abbia emanato, in un primo momento, un bando di gara in difformità di quanto previsto nella citata direttiva e che successivamente abbia proceduto alla stesura di un nuovo bando di gara. Allo stesso modo è stata dichiarata priva di fondamento l'asserzione che il bando stesso sia stato inficiato da «palesi e gravi errori di valutazione del servizio». È stato altresì riferito che il bando di gara ha previsto l'erogazione dei detti servizi, in particolare, quello relativo alla vigilanza, in tutte le scuole in cui tale attività è in atto e nel medesimo livello di erogazione del servizio stesso; ciò fatta eccezione per pochissime scuole, nei confronti delle quali, stanti alcune incongruenze di comunicazione, l'Ufficio ha provveduto alle indispensabili rettifiche riconoscendo alle scuole interessate le risorse necessarie. Con comunicazione inviata al Raggruppamento temporaneo di imprese aggiudicatario, Miorelli-Palmar, in data 2 luglio 2007, l'Ufficio ha definito gli importi contrattuali spettanti a ciascun istituto per le attività di vigilanza, in modo da consentire la sottoscrizione dei contratti attuativi presso le singole scuole, nel rispetto dei termini contrattuali. Soltanto per sei scuole della Regione, tra cui quattro scuole della Provincia di Lucca, è stato previsto un decremento del numero complessivo delle ore di vigilanza a seguito dì una specifica richiesta da parte dei rispettivi dirigenti scolastici, a fronte di una più attenta verifica delle esigenze organizzative e di servizio. Con riguardo al calcolo delle ore di vigilanza che sarebbero state decurtate, in particolare per le scuole della Provincia di Lucca il competente Ufficio scolastico regionale ha precisato che tale calcolo non è esatto considerando anche che in tutta la Regione il numero delle ore settimanali di vigilanza previsto, ivi comprese le scuole della Provincia di Lucca, ammonta a poco più di 6.000. Sulla questione si è svolto un confronto tra il Raggruppamento temporaneo di imprese aggiudicatario, le organizzazioni sindacali di settore e l'Ufficio scolastico regionale per quanto riguarda la problematica dell'assunzione dei lavoratori impegnati nel servizio. L'Ufficio ha fornito assicurazioni che il personale in servizio presso le ditte appaltatrici cessanti è stato assunto in carico dal Raggruppamento temporaneo di imprese aggiudicatario della gara. È stata segnalata, tuttavia, una situazione di difficoltà per quattro scuole della provincia di Lucca che l'Ufficio scolastico regionale sta verificando.

e, quindi, segnalava una realtà falsa o falsata; inoltre, il verbale del 9 maggio 2007, cui lei stesso fa riferimento, circa la salvaguardia dei livelli occupazionali, a partire dal 1° luglio

questione è la seguente. Questa impostazione contrasta, a nostro avviso, l'indirizzo del Governo e del Parlamento sulla necessità di procedere alla stabilizzazione dei lavoratori e delle lavoratrici precari ed è per questo motivo

a mio avviso fanno della gara al massimo ribasso un terreno insostenibile ed ingiusto che annulla i diritti dei lavoratori e la prospettiva di superare il precariato garantendo un lavoro stabile. Credo che il Ministero debba riflettere se in questi casi (tra l'altro anche in relazione alla normativa dei lavoratori ATA che dagli enti locali sono transitati transitati presso il Ministero) non sia opportuno escludere tassativamente forme di appalti al ribasso che non valorizzino la professionalità e l'efficienza dei servizi e soprattutto non tutelino i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori precari.

all'interrogazione presentata si ritiene opportuno anzitutto premettere che per la fornitura dei collegamenti ADSL non esiste alcun obbligo, né condizione di fornitura del servizio a carico degli operatori, in quanto i collegamenti a larga banda esulano dall'ambito del servizio universale, unica fattispecie per la quale possono essere imposti agli operatori obblighi del servizio. D'altra parte, è noto che il Ministero delle comunicazioni ha adottato ogni possibile iniziativa allo scopo di aumentare la diffusione di tale mezzo trasmissivo ed eliminare il cosiddetto *digital divide*, come dimostrano sia l'erogazione di contributi per i contratti di abbonamento al servizio di accesso a larga banda ad Internet, sia i finanziamenti previsti per gli investimenti effettuati dalla società Infratel. L'area di intervento, originariamente limitata al solo Mezzogiorno, è stata estesa a tutte le aree del Paese e con la legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono state ulteriormente incrementate le risorse specificamente destinate al finanziamento degli interventi di realizzazione delle infrastrutture per la larga banda e di completamento del programma di sviluppo della larga banda nel Mezzogiorno da parte del Ministero delle comunicazioni per il tramite della società Infratel Italia, prevedendo lo stanziamento di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, nonché l'assegnazione di ulteriori 50 milioni di euro per l'anno 2009 allo stesso Ministero delle comunicazioni per le suddette finalità. Allo stato, pertanto, la disponibilità totale dei fondi da parte della società Infratel è di 320,1 milioni di euro, dei quali, come sopra indicato, 80 milioni derivanti da stanziamenti previsti dalla legge finanziaria 2007. Va, inoltre, sottolineato che uno degli obiettivi di legislatura del Governo è proprio lo sviluppo della banda larga come nuova frontiera del servizio universale, come grande occasione di sviluppo del Paese e di alfabetizzazione tecnologica della popolazione. Per raggiungere tale risultato il Governo ha istituito nei mesi scorsi un Comitato della banda larga, di cui fanno parte, oltre al Ministro delle comunicazioni, anche il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali e il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, con lo scopo di coordinare, indirizzare e supportare tutte le attività finalizzate allo sviluppo della suddetta tecnologia nel territorio nazionale, a partire dall'approntamento di misure in grado di dare soluzione al problema del *digital divide*. Nel passato è mancato al nostro Paese un approccio strategico coerente a sostegno dello sviluppo del settore; il Comitato della banda larga è chiamato a colmare tale vuoto di iniziativa e ad elaborare una organica politica del Governo sul tema, in grado di raccogliere l'interesse e la condivisione di tutti i soggetti coinvolti, dalle amministrazioni locali agli operatori, dai fornitori di servizi agli utilizzatori, nella convinzione che solo operando in sinergia l'obiettivo potrà essere centrato. Ciò premesso in linea generale, per quanto concerne, in particolare, il comprensorio indicato nell'atto parlamentare, la società Infratel ha precisato che in effetti, ad esclusione del Comune di Roana (che è dotato di una infrastruttura abilitata a fornire servizi ADSL) gli altri centri non risultano coperti in larga banda, ma nel prosieguo del programma la stessa società Infratel potrebbe effettuare la copertura attraverso tecnologie *wireless*. Signor Presidente, devo dichiararmi insoddisfatto della risposta che oggi l'onorevole Sottosegretario ha voluto fornirci. L'Altopiano di Asiago, come noto, è un territorio di montagna con una vocazione principalmente dedicata al turismo e ai servizi e quindi con necessità di infrastrutture per consentire ai suoi abitanti di vivere, operare e creare ricchezza nel territorio. Oggi il servizio di trasmissione dei dati a banda larga - come ha riconosciuto lo stesso Sottosegretario - è uno strumento di *marketing* territoriale assolutamente indispensabile per sviluppare servizi sul territorio e dare risposte ai cittadini. Da ciò è nata l'esigenza di questa interrogazione a cui il Sottosegretario ha voluto rispondere. Quindi, ritengo assolutamente inaccettabile che le zone di montagna,

Tante volte, a parole, la politica dichiara di voler garantire alle popolazioni di montagna la possibilità di rimanere a lavorare nei propri territori e poi tutto sfocia in vuote dichiarazioni di principio. Nel concreto, troppi sono i disagi che le popolazioni di montagna devono ancora sopportare per continuare a vivere nei paesi di cui sono originari. L'interrogazione che chi parla ha presentato dimostra che talvolta, con modesti interventi ed investimenti, si potrebbero concretamente migliorare le condizioni di vita dei cittadini di montagna. Questo è ancor più vero per l'Altopiano di Asiago che da tempo lamenta una discriminazione a proprio danno di concorrenza sleale rispetto al trattamento dei vicini Comuni trentini, che per effetto di un ormai anacronistico Statuto di autonomia godono di privilegi assolutamente non compatibili e non comparabili con quelli dei Comuni veneti. Da qui la richiesta di adesione alle Province autonome di Trento e Bolzano, a cui i Media hanno dato ampio risalto. Per questo, onorevole Sottosegretario, non possiamo essere soddisfatti di una risposta così

all'ordine del giorno concernente le comunicazioni del Presidente sul contenuto del disegno di legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 126, commi 3 e 4, del Regolamento, Comunico che è pervenuto alla Presidenza il parere espresso dalla 5a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 126, commi 3 e 4, del Regolamento, sul disegno di legge n. 1817 che reca: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008)». Detto parere sarà pubblicato in allegato ai resoconti della seduta odierna. Tenuto conto del parere espresso dalla 5a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge finanziaria per il 2008, ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento, preso atto della posizione del Governo, comunico, in ordine al profilo dell'ambito contenutistico del disegno di legge finanziaria, che il testo presentato dal Governo, appare, nel complesso, in linea con le prescrizioni dell'articolo 11 della legge n. 468 del 1978 e successive modificazioni, tra cui da ultima la legge n. 208 del 1999, fatta eccezione per le seguenti disposizioni: - gli articoli 5,

e 80, in quanto violano il divieto di introdurre norme di carattere ordinamentale di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *i-bis),* della legge n. 468 del 1978 e successive modificazioni; gli articoli 4, commi da 23 a 26, 5, commi da 27 a 30,

articolo 17, in quanto, pur prevedendo un onere, presentano un contenuto non finalizzato direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia. come prescritto dall'articolo 11, comma 3, lettera *i-ter)*, della citata legge n. 468 del 1978 e successive modificazioni. Dispongo pertanto lo stralcio di tutte le citate disposizioni, che andranno a costituire autonomi disegni di legge.

alla 5a Commissione, in sede referente, con il parere di tutte le altre Commissioni permanenti e della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Le Commissioni sono pertanto sin da ora autorizzate ad integrare i propri ordini del giorno per l'esame di questi provvedimenti.

descrizione attenta, oltre che insindacabile, del documento di accoglimento da parte della Presidenza del Senato della relazione che la Commissione bilancio le ha fornito.

37, comma 2, possa veramente realizzarsi e non accada anche per la Regione Veneto quello che sta avvenendo per la Regione Sicilia, dove, a fronte di un provvedimento del tutto simile, ancora il Governo non ha costituito lo stanziamento necessario perché la società mista tra Regione e ANAS potesse espletare le proprie gare e procedure.